*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione di una «Giornata della memoria», emblematicamente il 9 ottobre, data della catastrofe del Vajont del 1963, è certamente condivisibile e lo è tanto più nella misura in cui rappresenti l'occasione di un serio approfondimento. La «Giornata Nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo» deve - a mio giudizio - indurre ad un'azione più costante, più attenta e più severa di tutela del territorio e dell'ambiente, di rigore nell'attività innanzitutto di prevenzione e poi di repressione dei reati ambientali, di attento monitoraggio delle aree industriali, con particolare riguardo agli scarichi e alle emissioni inquinanti l'acqua e l'aria, alla formazione di profili professionali specifici da indirizzare soprattutto verso gli enti locali, che spesso ne sono sprovvisti e - ciò che ciò che pregiudizialmente conta - ad una legislazione che colmi i vuoti e riordini la normativa vigente. A tale ultimo proposito, la prossima settimana in Commissione ambiente verrà incardinato un disegno di legge del quale sono primo firmatario, sottoscritto dalla presidente Finocchiaro e da tutti i senatori del Gruppo PD, in materia di «Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico», volto ad offrire un contributo nella direzione che ho appena indicato. Del resto, nel nostro Paese, da quel 1963 in avanti, si sono susseguiti nel tempo, e poi drammaticamente ravvicinati negli ultimi quindici anni, eventi calamitosi di varia entità, diffusi sull'intero territorio nazionale. Mi riferisco in particolar modo a violente alluvioni e fenomeni conseguenti al dissesto idrogeologico, alle esondazioni di corsi fluviali, ma la mente corre naturalmente, nella nella circostanza odierna, ai terremoti e ai disastri industriali. A tale ultimo riguardo, l'immane tragedia di Fukushima in Giappone e, sul territorio europeo, l'annuncio della Germania di una decisa inversione di tendenza nell'approccio al tema del nucleare sul proprio territorio nazionale, postulano interrogativi ai quali il quesito referendario, proprio oggi validato dal pronunciamento della Corte di cassazione, che disillude definitivamente le aspettative del Governo, potrà dare adeguata risposta grazie all'auspicato consenso del corpo elettorale. Quando si parla di disastri ambientali è fatale che ciascuno di noi si riferisca a drammatici eventi che hanno segnato il proprio territorio: territorio: penso a Sarno, all'alluvione del 1998 che coinvolse anche i comuni di Siano e di Bracigliano, anch'essi in provincia di Salerno, ed ancora Quindici, San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Ero in quel momento, e già da qualche anno, Presidente della Provincia di Salerno, un territorio che qualche decennio prima, nel 1954, era stato colpito da una violenta alluvione che aveva mietuto numerosissime vittime. Ma Sarno è, per certi versi, drammaticamente "intonato" al tema di oggi, perché nel titolo del disegno di legge in esame si parla di incuria dell'uomo. Certo, non si può dire diversamente - me ne rendo conto - ma occorrerebbero ben altri sostantivi, seguiti da aggettivi altrettanto espliciti, per definire talune situazioni. A Sarno, nel 1998, 137 morti (poi, 6 a Bracigliano e 5 a Siano, per restare al solo contesto salernitano). Tra questi, interi nuclei familiari sterminati! In un vallone, che normalmente avrebbe dovuto assolvere al compito di canalizzare l'acqua piovana, i detriti della montagna in caso di smottamenti (pietriccio, materiali piroclastici e del sottobosco, fango, alberature)

Si tratta di quattro opere pubbliche: una scuola materna, una biblioteca comunale, un centro sociale ed una palestra comunale, nella quale furono poi allineate le bare via via che venivano scavati dal fango e dalle rovine delle case crollate i corpi delle vittime. Quei quattro edifici, ostruendo il vallone, certamente provocarono una deviazione del corso dei materiali franosi, che perciò investirono l'abitato, determinando un numero - a mio avviso - ancora maggiore di vittime rispetto a quello già elevato che l'alluvione avrebbe prodotto. Sono ancora presenti dinanzi agli occhi di tanti di noi le immagini del disastro provocato dal torrente Dragone ad Atrani, in costiera amalfitana, il 9 settembre dello scorso anno. Dopo giorni e giorni, il corpo di Francesca Mansi fu trovato al largo di Lipari: un'altra vita spezzata, per giunta in così giovane età, un'altra povera vittima dell'«incuria dell'uomo», appunto. Questi tragici bilanci non vorremmo registrarli mai più. Di qui scaturisce la necessità non solo di ricordare, ma - come giustamente il relatore, collega Bianco, afferma - anche di informare, di sensibilizzare nella giornata dedicata e - io aggiungo, certo di incontrare la condivisione unanime di quest'Aula - di utilizzare quel giorno e tutti gli altri dell'anno e degli anni a venire per operare in difesa del territorio, per mettere in sicurezza l'abitato, per liberare le aree a rischio elevato, delocalizzando quanto c'è da delocalizzare, investendo per questo risorse vere, pur nella consapevolezza della incontenibile necessità, sotto il profilo finanziario, per far fronte a fenomeni così particolari e diffusi. Come pure, signor Presidente, appare necessario prestare maggiore attenzione al tema dei risarcimenti alle famiglie delle vittime, assicurando assoluta tempestività per alleggerire almeno i risvolti materiali dei disastri. Anche qui cito un esempio della mia terra: a Nocera Inferiore, il Comitato vittime della frana che ebbe in luogo in località Starza il 4 marzo del 2005 ancora si adopera, ma senza successo, affinché siano erogati sono trascorsi ormai 6 anni - i risarcimenti agli aventi causa. Mentre si celebra, proprio quest'anno, l'Anno europeo del volontariato, mi pare doveroso, nel rivolgere un pensiero a tutte le vittime dei disastri ambientali e industriali, inchinarmi di fronte anche a quell'autentico pacifico esercito di volontari che in questo Paese interpreta un ruolo assolutamente insostituibile, che anzi in passato - in fondo in un passato recente - fu capace di supplire alle troppe negligenze e deficienze dei sistemi di emergenza e di una Protezione civile che ancora stentava a prendere forma e ad essere culturalmente e funzionalmente assunta dalle istituzioni italiane.

determinano quindi gravissimi danni, non solo alle persone, ma anche ai centri abitati, alle infrastrutture e ai nostri beni ambientali, storici e culturali. In Italia sono state recentemente censite dall'ISPRA e delle Regioni oltre 485.000 frane,

Quasi mai, però, i danni e le vittime sono causati direttamente da fattori ambientali. Anzi, molto spesso la vera causa di questi problemi è costituita dal mancato rispetto, dalla mancata osservanza delle regole tecniche e dei vincoli di natura legislativa o amministrativa.

la commemorazione delle vittime di queste situazioni. Però io credo che, partendo da questo provvedimento, noi dobbiamo sollecitare e attenzionare il nostro interesse e il nostro impegno affinché si abbia una continua e puntuale applicazione delle leggi (ovviamente aggiornandole, laddove ciò sia ritenuto opportuno) e vi sia un continuo monitoraggio di tutti i mezzi di ispezione e prevenzione volti ad evitare questi disastri. Il Gruppo dell'Italia dei Valori è stato sempre molto attento a questi temi. Abbiamo presentato diverse mozioni, disegni di legge ed anche emendamenti

le nobili finalità del testo di questa iniziativa legislativa. Credo tuttavia - come ho già detto - che occorra pensare a nuovi strumenti e soprattutto a risorse che ci consentano di evitare i disastri che sono accaduti

che, intervenendo sulla prescrizione dei reati, renderebbero praticamente inapplicabili le sanzioni oggi vigenti in materia di edilizia, di urbanistica e di paesaggistica, dal momento che quasi tutta la legislazione in materia ambientale è imperniata su un quadro sanzionatorio di tipo amministrativo. Auspichiamo che questi provvedimenti continuino a giacere lì dove si trovano e non vedano mai la luce. D'altra parte rileviamo anche che molti Paesi europei hanno una legislazione molto più avanzata della nostra, anche in materia di delitti ambientali. Il nostro

la discussione che oggi si svolge in Aula possa essere di stimolo per tutti noi per avviare una seria ed approfondita ricognizione dello stato del nostro territorio e soprattutto una vera

La storia di queste comunità venne sconvolta dalla costruzione della diga del Vajont, che determinò la frana del monte Toc nel lago artificiale. La sera del 9 ottobre 1963 si elevò un immane ondata, che seminò ovunque morte e desolazione. La frana che si staccò alle ore 22,39 dalle pendici settentrionali del monte Toc, precipitando nel bacino artificiale sottostante, aveva dimensioni gigantesche. Una massa compatta di oltre 270 milioni di metri cubi di rocce e detriti fu trasportata a valle in un attimo, accompagnata da un'enorme boato, provocando oltre 2.000 vittime. Fu aperta un'inchiesta giudiziaria. Il processo venne celebrato, nelle sue tre fasi, dal 25 novembre 1968 al 25 marzo 1971 e si concluse con il riconoscimento di responsabilità penale per la prevedibilità di inondazione e di frana e per gli omicidi colposi plurimi. Il 9 ottobre 2008 vengono portati a Longarone e resi disponibili gli atti

Non dimentichiamo che la provincia di Belluno è stata in passato, fin dall'800, terra di grande emigrazione per difficoltà di lavoro e che proprio in quegli anni la ripresa economica e lo sviluppo avevano dato i primi segnali di controtendenza. La zona in cui si è verificato l'evento catastrofico continua a parlare alla coscienza di quanti la visitano attraverso la lezione, quanto mai attuale, che da esso si può apprendere. Ringrazio quindi il Parlamento che vuole dimostrare profonda sensibilità e vicinanza ai discendenti e a quella terra. Non sono però pienamente soddisfatto del titolo del disegno di legge, in particolare della parola "incuria", come è stato rappresentato anche dai sindaci dei comuni di Erto e Casso, Vajont, Castellavazzo e Longarone;

Altre sono riconosciute come catastrofi ambientali causate da questa negatività di comportamento dell'uomo. In assoluto, potremmo dire che il male peggiore ovviamente è la guerra.

Vorrei ricordare il disastro dovuto alla piattaforma della BP, la Deepwater Horizon, nelle acque del Golfo del Messico, oppure ancora il disastro causato dall'impianto nucleare giapponese di Fukushima. l'uomo, il genere umano, sta raggiungendo capacità di spostare materiali più di quanto il pianeta faccia con imprese naturali di sedimentazione, di orogenesi e di dinamica delle placche. L'uomo sta diventando una forza della natura che ha impatti devastanti sulla stessa Terra. Forse si può anche pensare a nuove generazioni di geoesperti, in modo di comprendere meglio i processi che hanno modellato l'ambiente terrestre, per preservarlo e per tramandarlo alle future generazioni, integro come ci è stato consegnato.

con il quale, proprio per dare sostanza a questa Giornata di memoria, chiediamo che presso il Ministero dell'interno sia previsto uno speciale Fondo per finanziare progetti di gestione e manutenzione del sacrario delle vittime del disastro del Vajont

Signor Presidente, il mio è un intervento per illustrare l'ordine del giorno G1. Comunque anch'io colgo l'occasione del dibattito sul disegno di legge che istituisce la Giornata in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali per ricordare una delle tragedie più gravi successe nel nostro Paese, di cui già hanno parlato alcuni colleghi. Mi riferisco in particolare al disastro del Vajont

quel disastro, come tanti altri che si sono susseguiti nel nostro Paese, sono stati provocati non solamente dall'incuria dell'uomo, ma sono stati causati da comportamenti omissivi o attivi dell'uomo. Proprio per quanto riguarda il Vajont, come è già stato detto, si è trattato di una immensa frana che è andata ad impattare

che hanno provocato tale disastro: un disastro preannunciato, un disastro che si poteva evitare.

che è stata documentata in una ricca bibliografia, in testi, libri, film, rappresentazioni teatrali, ma è stata anche oggetto di ricerca e d'indagine di università italiane e internazionali. Sta di fatto che in quella occasione è stato privilegiato il progetto della società SADE, insieme all'ENEL, per costruire la diga più alta del Paese e l'impianto idroelettrico idroelettrico più imponente. Non si è voluto ascoltare e vedere. Non si è voluto ascoltare alcuni esperti e la popolazione, che con preoccupazione andava in piazza anche quando si lavorava alla nuova diga. Non hanno voluto vedere le piccole frane e le crepe sulle strade e sugli edifici. Vorrei ricordare che a ridosso dell'evento una giornalista de «l'Unità», Tina Merlin, ha scritto con preoccupazione, ma anche con dettagli della consapevolezza che qualcosa doveva succedere.

in maniera sufficiente le vittime, i danni morali e materiali di quella popolazione e di quel territorio, come anche le vittime degli altri disastri del nostro Paese, però ciò non ci esime dal ribadire - questo cerco di farlo anche con l'ordine del giorno G1 che porta la mia prima firma - e rafforzare l'impegno di noi tutti, del Governo *in primis* e delle autonomie locali, affinché vengano posti in essere tutti gli atti e tutte le azioni per prevenire tali disastri,

comportamenti ed interventi assolutamente aggressivi sulla natura e sul paesaggio. Si tratta di temi molto attuali anche oggi, ai quali bisogna dare delle risposte. Nel sostenere l'ordine del giorno G1, voglio ricordare anche io che le Nazioni Unite nel febbraio del 2008, all'Assemblea generale per presentare il giorno internazionale del pianeta terra, hanno citato il disastro del Vajont assieme ad altri quattro come esempio di disastro evitabile, causato dalla scarsa comprensione delle scienze della terra

la legge che oggi verrà approvata, insieme agli ordini del giorno presentati, che vanno in qualche modo ad arricchire il testo della legge, possa veramente servire affinché queste cose non si ripetano.

per osservare che il disegno di legge è anche, e forse soprattutto, una sorta di tributo del Parlamento italiano alla memoria di popolazioni, famiglie e cittadini che sono stati duramente colpiti, come altri colleghi hanno ricordato, il 9 ottobre del 1963. Ebbene, questo tributo alla memoria purtroppo non è perfettamente riuscito. Il Parlamento istituisce una giornata in memoria delle vittime dei disastri causati dall'incuria dell'uomo partendo da una sciagura, quella del Vajont, che non fu determinata dell'incuria degli uomini, ma da comportamenti colpevoli e delittuosi, comportamenti di uomini che anteposero la logica del profitto e di un malinteso sviluppo alla doverosa tutela del territorio, delle popolazioni e delle vite umane. È grave, signor Presidente, colleghi, che dopo quasi cinquant'anni da quella giornata così tragica

È evidente che noi oggi istituiamo una giornata che non fa riferimento soltanto alla tragedia del Vajont, ma da quella tragedia partiamo, e non usiamo le parole giuste: in qualche modo, torniamo inconsapevolmente a ferire le popolazioni che coltivano la memoria di quel tragico evento. Quando si parla di memoria e di ferite ancora aperte, anche le parole andrebbero pesate meglio. In questo senso, signor Presidente,

Vaccari, che affrontano tale problema, ancora così sentito. Non ho altro da aggiungere alle parole che altri colleghi hanno pronunciato in quest'Aula, ma voglio soltanto sottolineare che questa è l'occasione per inchinarci una volta di più alla memoria delle vittime, dei loro familiari e per impegnarci tutti affinché

sono stati causati da gravi errori dell'uomo, ribadisce che nel titolo e nell'articolato del disegno di legge il termine incuria va inteso e comprende anche i comportamenti attivi od omissivi di particolare gravità e non solo di semplice noncuranza, negligenza o disattenzione».

Il Governo concorda perciò pienamente con la proposta del relatore e ringrazia per la disponibilità i colleghi che hanno trasformato in ordine del giorno l'emendamento.

l'Italia dei Valori voterà a favore di un disegno di legge che richiama tutti alla lezione della memoria: la memoria di eventi dolorosi del passato, ma anche della scelta di fondo che la politica e le istituzioni debbono operare su come porsi in rapporto con i cittadini. Una tra le tante possibili lezioni che viene dal voto amministrativo recente, confortata da un'analisi della legislazione industriale e ambientale degli ultimi decenni, è che l'obiettivo della crescita non è disgiungibile dal rispetto del territorio e che il rispetto del territorio è è possibile solo se si ascoltano i cittadini e le rappresentanze elettive territoriali. Se queste ultime non svolgono il proprio compito, o se qualcuno specula illecitamente sul territorio e danneggia l'ambiente, allora entra in gioco il ruolo dello Stato nel predisporre una legislazione efficace, efficiente e puntuale a tutela del bene ambiente. Se i Comuni, la magistratura e le forze dell'ordine vedono ridotte le proprie risorse, se i tagli trasversali, orizzontali e indiscriminati colpiscono anzitutto gli organismi che sul territorio devono svolgere il controllo e il monitoraggio sulle opere e sulle modalità di spesa, allora ci troveremo sempre a commemorare vittime di eventi che, per dirla con Ciampi, «potevano e dovevano essere evitati». Il moltiplicarsi delle commemorazioni ha un senso solo se si accompagna a politiche efficaci. I dati sul dissesto idrogeologico, sulla fragilità del suolo, sulle frane e le alluvioni sono noti. Non sono, invece, altrettanto noti i dati su come siano stati spesi i soldi per prevenire il rischio idrogeologico e sismico, su quali interventi siano stati cantierati e quanti siano stati ultimati, su cosa abbiano fatto i commissari straordinari che l'ultima legge ha creato. Questi elementi abbiamo chiesto di conoscere con gli ordini del giorno G2 e G3 - riferiti al rapporto tra attività umane ed ambiente - visto che l'elemento della consapevolezza è valorizzato proprio dal disegno di legge in esame e che senza innovative politiche di prevenzione l'incuria continuerà a produrre disastri come quelli, piccoli e grandi, che si sono moltiplicati dopo il Vajont. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo dell'UDC-SVP e Autonomie sul testo alla nostra attenzione. Si tratta di un provvedimento approvato a larghissima maggioranza dall'altro ramo del Parlamento di un fenomeno che ci preoccupa tutti, sia per quanto riguarda il passato, al quale dedichiamo la giornata della memoria, ma anche per le preoccupazioni che si rivolgono al futuro.

In relazione alla storia italiana il pensiero non può che andare, *in primis*, alla tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963,

ed ambientali, ma anche nell'impegno che, con l'approvazione del provvedimento, l'Italia assumerebbe a organizzare iniziative tese a ricordare il rispetto per il patrimonio ambientale e le conseguenze derivanti da un suo deterioramento, nonché momenti di riflessione sul rapporto tra sviluppo e tutela ambientale. Un rapporto sempre in tensione che ci dovrebbe far riflettere, anche per quanto riguarda l'energia nucleare, e sul quale dobbiamo, per fortuna, grazie alla Corte di Cassazione, decidere il 12 e il 13 giugno. Come Come risulta da recenti indagini, condotte in particolare da Legambiente e dal Dipartimento della Protezione civile con Ecosistema Rischio 2010, l'Italia si scopre purtroppo sempre più fragile, non solo per la forte presenza di aree ad alta criticità idrogeologica - condizione che caratterizza ben 6633 comuni - ma anche per il grave ritardo nelle attività di prevenzione. Ricordo i seguenti dati. Nell'82 per cento dei comuni intervistati da Ecosistema rischio 2010 sono presenti abitazioni in aree golenali, in prossimità degli alvei e in aree a rischio frana, dei casi non sono singole case, ma addirittura interi quartieri. Nel 54 per cento delle municipalità sono presenti, in aree esposte al pericolo di frane ed alluvioni, fabbricati industriali per cento, strutture pubbliche sensibili, come scuole e ospedali. Complessivamente, si può stimare che ogni giorno nel Paese siano oltre 3 milioni e 500.000 i cittadini esposti al pericolo di frane e alluvioni. Considerata la delicata e preoccupante situazione, è quindi necessaria una concreta politica di prevenzione attraverso la quale affermare una nuova cultura del suolo e del suo utilizzo, per non assistere mai più a drammatiche vicende quali quelle avvenute in passato. Colgo, inoltre, l'occasione che ci offre l'auspicata approvazione di queste norme di civiltà, e in special modo l'introduzione di questa giornata della memoria, per porre all'attenzione dell'Assemblea una richiesta diversa sollevata più volte, e in più occasioni, da tanti senatori su un tema altrettanto importante, quale il ripristino degli effetti civili di alcune festività religiose. Lo sottolineo perché in questa Aula ci sono stati tanti interventi in questo senso. Il primo era quello (non è ora presente ma lo vorrei ricordare) del senatore Cosimo Izzo, che già nel 2001 aveva presentato un disegno di legge sottoscritto da 160 senatori. tutto rimasto nel cassetto. Io stesso ho presentato nel 2001, ripresentandoli nel 2006 e nel 2008, vari disegni di legge per salvare almeno una di queste festività abolite. Sono iniziative da considerarsi favorevolmente alla luce del fatto che appartengono alla nostra cultura, al patrimonio religioso di tanti cittadini oltre che alla nostra storia. Nella Nella consapevolezza, da un lato, di rendere ossequio alle vittime dei disastri ambientali e industriali e, dall'altro, di dare risposta alla necessità sempre più urgente di iniziative volte a promuovere una sensibilizzazione verso il valore del rispetto e della tutela del territorio, nonché di affermare una nuova cultura del suolo e del suo utilizzo, il Gruppo dell'Unione di Centro, SVP e Autonomie esprimerà pertanto convintamente il proprio voto favorevole al provvedimento al vaglio dell'Assemblea e dunque all'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri

al cospetto di tragiche calamità è il doloroso sconcerto nel constatare l'incapacità di trarre profitto dalle sciagure del passato. Troppo sovente pare che la cosiddetta cultura dell'emergenza si riduca all'adeguatezza dell'intervento nella situazione contingente. Si confida, cioè, nella generosa efficienza di corpi professionali o di volontari, dai Vigili del fuoco alla Protezione civile (per citare solo due tra le numerose istituzioni benemerite), mentre appare ancora insufficiente l'attenzione dedicata al capitolo della prevenzione e, dunque, della responsabilità. Credo che questa constatazione racchiuda il senso più profondo del disegno di legge volto a istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo. Doverosa la rimembranza delle vittime, ma non meno indispensabile è che di tante tragedie si faccia tesoro affinché simili sciagure non abbiano più a verificarsi. I 2.000 morti del Vajont, che altri colleghi hanno ricordato, nell'immane disgrazia che ha segnato in maniera indelebile la nostra memoria collettiva e che ora si pone a pietra miliare del ricordo, non sono frutto di crudele fatalità, bensì della violenza operata sull'ambiente, e soprattutto il funesto esito di scelte sconsiderate che comportano rischi gravissimi per l'intera comunità. Comprensibile, dunque, che a qualcuno appaia blanda la definizione di incuria dell'uomo, come ben ha fatto il senatore Vaccari, impiegata nel disegno di legge per classificare la causa di avvenimenti talmente funesti. Tuttavia, eccezion fatta per episodi determinati da un dolo evidente e volontario (e di ben minore entità, come le devastazioni causate da piromani), le esperienze passate dimostrano come a giocare un ruolo determinante nelle più luttuose circostanze sia precisamente l'irresponsabile noncuranza rispetto a un potenziale pericolo collettivo. Da qui, l'importanza di un provvedimento quale il presente che, all'articolo 2, esprime la propria finalità nel promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio. In questa opera di formazione delle coscienze la cattedra più alta spetta alle vittime delle sciagure e rileviamo con soddisfazione l'opportuna scelta di sposare la celebrazione della memoria all'opera di sensibilizzazione. Per parte nostra abbiamo chiesto che, nell'approssimarsi della cinquantesima ricorrenza del disastro del Vajont, si provveda anche a contribuire adeguatamente alle esigenze di gestione e manutenzione del sacrario delle vittime di quel tragico 9 ottobre 1963. Facciamoci carico fino in fondo, colleghi senatori, del debito collettivo assunto nei confronti di cittadini a cui lo Stato non ha saputo garantire la prima delle prerogative: il diritto all'incolumità e alla vita.

dei deputati. Pertanto, il prossimo 9 ottobre - anche se auspico che ciò non accada solamente nella giornata del 9 ottobre ma diventi prassi quotidiana - avremo modo di dedicare alcune iniziative per ricordare le vittime dei disastri ambientali ed industriali ma soprattutto per promuovere una nuova cultura, una nuova consapevolezza una sensibilizzazione sui temi che oggi abbiamo trattato in questa sede, che riguardano la sicurezza e l'incolumità delle persone, nonché il giusto equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale. Ritengo che un Paese civile non possa più permettere che avvengano disastri come quello del Vajont e simili. Sono temi - come ho già avuto modo di dire poc'anzi - di grande attualità, che in qualche modo mettono in discussione i

che hanno espresso alcune perplessità sul termine usato nel titolo di questo disegno di legge. Mi auguro che gli ordini del giorno accolti possano soddisfare le loro richieste. Anch'io vorrei ringraziare i colleghi della I Commissione della Camera, l'onorevole Rossa, prima firmataria del disegno di legge, i colleghi della 1a Commissione del Senato e il relatore, senatore Bianco. Non mi resta dunque a nome del Gruppo del Partito Democratico, il voto favorevole sul disegno di legge.

Signor Presidente, in questo scorcio di terzo millennio è sempre più condivisa la necessità di pervenire ad un nuovo approccio alla disabilità, passando dal cosiddetto modello medico al cosiddetto modello sociale. Per modello medico si intende un approccio che mette in primo piano le menomazioni e la persona in secondo piano. Al contrario, l'approccio basato sui diritti promuove un cambiamento di valori e un abbandono di questo modello a favore di un modello sociale, che considera la persona con disabilità come soggetto attivo di diritti e non come oggetto passivo di assistenza. Conseguenza logica di tale approccio è la consapevolezza che l'accesso ai diritti fondamentali, come la salute, la riabilitazione o l'educazione permanente, non può essere negato a nessuno sulla base della disabilità o di altre condizioni, inclusa l'età. In questa prospettiva i sistemi sanitario, di protezione sociale e scolastico non possono, per nessuna ragione, limitare o violare alcun diritto individuale riconosciuto dalle normative internazionali e nazionali. L'accesso a programmi di riabilitazione e all'istruzione dovrebbe essere, quindi, riconosciuto come una priorità e garantito a tutti, indipendentemente dal tipo di disabilità. Sono delle difficoltà finanziarie, ma l'articolo 32 della Costituzione definisce la salute quale diritto fondamentale dell'individuo. È riconosciuto che i disturbi dello spettro autistico determinano una disabilità significativa, che perdura per tutta la vita. A causa della complessità dei loro bisogni, le persone con autismo formano un gruppo molto vulnerabile anche tra gli individui con disabilità. Ciò nonostante, non dovrebbero essere considerate o trattate come un'eccezione tra le disabilità e nemmeno come una popolazione che non è in grado di conseguire obiettivi quali l'indipendenza, l'autodeterminazione e la dignità. Queste persone hanno un valore umano immenso.

delle persone con autismo nelle aree deficitarie della comunicazione, delle capacità cognitive e del comportamento adattivo. Tuttavia, il supporto necessario a queste persone si traduce essenzialmente in termini di conoscenze e competenze specifiche di tutti gli attori coinvolti nell'intervento, e in particolare competenze specifiche del personale sanitario nel campo della diagnosi, valutazione e trattamento, informazioni corrette e accessibili alle persone interessate o ai genitori di coloro che sono incapaci incapaci di rappresentarsi da soli, sulle condizioni, sui bisogni generali e individuali delle persone con autismo e sui piani individualizzati di trattamento; adattamento ragionevole dell'ambiente al fine di favorire l'inclusione sociale e la piena partecipazione delle persone con autismo; competenze del personale incaricato di supportare le persone con autismo in ogni situazione di vita, comprese le attività lavorative e ricreative. L'assenza di questo tipo di supporto genera ulteriore disabilità, impedendo loro di realizzare il proprio potenziale individuale e di conseguire il maggior grado possibile di indipendenza, come pure la capacità di fare scelte responsabili e di autorappresentarsi, elementi chiave per assicurare dignità di vita e piena partecipazione. Un intervento sanitario ed educativo carente ha un impatto non solo su queste persone, ma anche su quelle coinvolte insieme a loro, e in particolare sulle famiglie, su cui, in caso di latitanza delle istituzioni, viene esercitata una pressione sproporzionata. Inoltre, a causa della normale aspettativa di vita delle persone con autismo, il futuro che le attende quando i loro genitori sono troppo anziani, malati o addirittura defunti rappresenta una grande preoccupazione per le famiglie. Un *network* di servizi che garantisca la continuità e qualità di cure necessarie per vivere una vita adulta dignitosa fornisce anche il più efficace sostegno emotivo alle famiglie. Non dobbiamo lasciarli soli. L'autismo, in particolare, è ormai considerato, secondo le indicazioni consolidate della letteratura internazionale, come una patologia precoce del sistema nervoso centrale che determina poi una disabilità complessa che colpisce pervasivamente la comunicazione, la socializzazione ed il comportamento. La causa o le cause precise non sono ancora note. A tutt'oggi l'autismo non è diagnosticabile alla nascita, perché viene identificato attraverso modelli di comportamento che si manifestano nel bambino dai 18 mesi ai 3 anni. A volte si assiste a periodi di sviluppo che apparentemente sono normali, dopo i quali il bambino sembra regredire e perdere le proprie capacità. Non c'è una vera e propria spiegazione esauriente a tutto ciò, e ovviamente questo comporta un senso di angoscia e di confusione nelle famiglie, spesso accusate di essere responsabili del deterioramento del proprio figlio. Ora sappiamo, invece, che i genitori sono la risorsa più importante per il bambino. Non appena si presentano le prime difficoltà, le famiglie necessitano di sostegno per la cura dei figli. Una diagnosi precoce, seguita da un trattamento educativo precoce, può aiutare a prevenire l'insorgenza di molte conseguenze secondarie di questo disturbo (quali ansia cronica, fobie e comportamenti difficili) e favorire l'apprendimento e lo sviluppo del bambino. I genitori dei bambini autistici hanno apportato un notevole contributo alla creazione di servizi - li ringrazio personalmente, perché ho vissuto con loro momenti davvero toccanti - e alla promozione e comprensione a livello mondiale, oltre ad essere rappresentati in alcune delle più importanti iniziative di ricerca concernenti tale disturbo. I bambini autistici diventano adulti con autismo e, sebbene un'educazione ed una presa in carico adeguata possano rappresentare un'enorme differenza nella loro capacità di affrontare la vita, i problemi sottostanti persistono. Gli studi condotti negli Stati Uniti, ma anche in Europa, nell'ultimo decennio, riportano un generalizzato aumento delle diagnosi di autismo, con una prevalenza fino a 8 su 1.000 del complesso dei disturbi dello spettro autistico (è fonte dell'Istituto superiore di sanità del 2009), la letteratura internazionale stima la nascita di un bambino con disturbi dello spettro autistico ogni 150 nati, con i maschi colpiti 4 volte più delle femmine.

Come si vede, i dati che abbiamo riferito sottolineano ancora una volta la presenza di servizi a macchia di leopardo sparsi sul territorio nazionale. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ricordo che 1'11 ottobre del 2010 l'Istituto superiore di sanità, nel corso di un convegno, ha annunciato la partenza nel 2011 di un progetto Certamente, a fronte di tale annuncio, desta non poca preoccupazione la scarsità di fondi a disposizione per la ricerca stessa. Come in tutti i settori, ma in questo maggiormente, occorre sviluppare diverse direzioni di ricerca per colmare rapidamente il vuoto di conoscenze sulle basi neurobiologiche di detti disturbi. Un impegno in questa direzione potrebbe favorire l'individuazione di potenziali terapie, possibilmente applicabili, in fasi precoci dello sviluppo, e mirate a migliorare la qualità della vita dei bambini autistici e dei loro familiari. Per quanto riguarda la necessità di una tempestiva diagnosi, è di tutta evidenza che quanto più questa viene effettuata tardivamente ben oltre il terzo anno di età - tanto più ciò comporterà un ritardo degli interventi terapeutici, a cui si associa una prognosi meno favorevole. L'efficacia degli interventi terapeutici aumenta se essi sono iniziati precocemente durante lo sviluppo del bambino. In tal senso andrebbe aumentata la consapevolezza degli operatori della scuola dell'infanzia e primaria; andrebbero maggiormente coinvolti anche i pediatri di base a livello locale,

di promuovere, con adeguati finanziamenti, anche in collaborazione con l'università, la ricerca nei vari aspetti; di adottare provvedimenti di carattere generale che impegnino le Regioni a definire modelli organizzativi

con le Regioni, un registro di prevalenza dei disturbi dello spettro autistico; a promuovere forme di coordinamento e collaborazione tra le istituzioni interessate al fine di sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale delle persone con autismo;

Colleghi, impegniamoci affinché la vita di una persona autistica diventi appagante e felice come quella di chiunque altro.

una patologia che deve ancora essere studiata attentamente; alcuni hanno individuato delle alterazioni dei neuroni, ma ciò non è ancora confermato. Si tratta di una patologia in aumento: questo appare chiaramente dalle certificazioni relative

se intervenga o meno un altro fattore, oltre a quello genetico e comportamentale. Sono stati documentati, associati a questa patologia, dei disturbi gastrointestinali con lesioni dei villi. Si tratta quindi

stabilire finalmente delle linee guida ben precise per i pazienti: le linee guida sono complesse e pregnanti nel caso di questa malattia, perché significano non una pastiglia o una terapia per qualche anno, ma la presa in carico globale della persona e della sua famiglia

inoltre utile passare dal gruppo di studio, che ha lavorato su questa malattia e che ha già proposto delle soluzioni, ad un *forum* nazionale per l'autismo, nonché porre molta attenzione

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, cosa fa il nostro Paese per i suoi cittadini che hanno disturbi dello spettro autistico? Li conosce? Sa della complessità della loro vita? È sulle risposte a queste domande che si concentra oggi l'attenzione dell'Aula del Senato, grazie alla mozione, a prima firma della al nostro esame, che intende impegnare il Governo, ma direi la Repubblica, affinché i diritti di cittadinanza non vengano mai meno, anzi siano rafforzati nei percorsi di vita che presentano problemi tra i più difficili da affrontare. Troppa è ancora la distanza tra le difficoltà che i disturbi dell'autismo comportano e le risposte scientifiche, sanitarie e sociali che oggi vengono offerte, tra il diritto all'autonomia, diciamo pure alla libertà, all'inclusione sociale e lavorativa, alla partecipazione, e la dipendenza che invece solitamente registriamo. In Italia si può e si deve fare di più. Questo innanzitutto è ciò che vogliamo dire oggi. Si può fare di più sul piano della ricerca, sulla quale è fondamentale investire, anche in vista di una qualche forma di prevenzione. Si può fare di più sulla specializzazione, capillare, dei medici, sia della fascia pediatrico-adolescenziale sia dell'età adulta, perché i problemi dell'autismo non finiscono a 18 anni, ma continuano. Si può fare di più sui percorsi scolastici e su quelli lavorativi, sull'organizzazione degli spazi di vita, in casa e fuori, nei luoghi pubblici ed in quelli di vacanza, sulle relazioni sociali. Si può fare di più sul sostegno alle famiglie, spesso in solitudine di fronte al problema, costrette a spese elevate, vittime di illusioni. Si può fare di più sull'informazione, perché l'opinione pubblica sia consapevole. Si può fare di più sulla formazione degli operatori. I disturbi dell'autismo da anni sono studiati dagli organismi internazionali della sanità e dai centri di ricerca. Vogliamo che l'Italia ne sia partecipe in modo più robusto e vogliamo che sia assicurata in tutto il territorio nazionale una rete di servizi, osservatori, centri diagnostici e assistenziali, che integri i servizi sanitari, la scuola, i percorsi sociali e lavorativi, in modo che sia data sicurezza alle famiglie, facendo sentire al loro fianco le strutture pubbliche e l'intera società. Noi oggi possiamo e dobbiamo dare indicazioni precise al Governo per un impegno che consenta di fare passi avanti sulla strada che pure si è aperta in questi anni. Il Tavolo nazionale di lavoro sull'autismo, che nel febbraio 2008 ha presentato la sua relazione finale, ricca di indicazioni, può concludere l'elaborazione delle linee-guida, che auspichiamo possano essere emanate al più presto. È necessaria una strategia nazionale, fondata sulla integrazione delle politiche di tutti i Ministeri interessati (cito il Ministero della salute e quelli dell'istruzione, del lavoro, degli affari sociali), ed è al contempo necessario un coordinamento forte tra le Regioni perché in tutto il territorio nazionale si sviluppino programmi integrati. Ricordo che dal 2002 la Regione Marche e dal 2004 la Regione Emilia-Romagna hanno adottato linee-guide, emanando direttive alle ASL, ma ad oggi solo la metà delle Regioni lo ha fatto. Occorre investire risorse: le ultime (500.000 euro) risalgono al 2007. Si tratta della vita delle persone. Si tratta di numeri non irrilevanti e crescenti. Un luogo strategico dell'impegno delle strutture pubbliche è, come è noto, costituito dalla scuola, a partire da quella dell'infanzia: una scuola di tutti a misura di ciascuno, anche per i ragazzi autistici. La Costituzione vuol dire questo: essi non sono ai margini ma nel cuore della visione costituzionale. Già il Consiglio europeo dei diritti sociali, in materia di educazione degli alunni autistici, ha dichiarato in una sentenza che l'educazione non è tale se non è efficace: l'efficacia come principio democratico, che afferma la corrispondenza tra diritti e risultati. Per questo esistono i Parlamenti ed i Governi. Per questo si battono i cittadini: semplicemente per questo, perché ai diritti corrispondano i risultati. Se partiamo dalle esperienze dei ragazzi, di tutti i ragazzi, è chiaro che il numero eccessivo di alunni per classe, la diminuzione dei docenti e la loro precarietà, l'assenza o la discontinuità dell'insegnante di sostegno, la frammentazione dell'organizzazione scolastica, la diminuzione del tempo-scuola, che i tagli colossali operati dal Governo hanno determinato in questi anni, mettono ostacoli al diritto all'istruzione, fino a vanificarlo. E questo vale per tutti e, soprattutto, per i ragazzi più deboli, come i ragazzi autistici, che hanno bisogno di attenzione, di relazione con gli altri, di tempo, di percorsi personalizzati; hanno bisogno della stabilità dei docenti. La recente proposta legislativa di privatizzare l'area del sostegno nella scuola non potrebbe che peggiorare lo stato delle cose, così come deve essere chiaro che bisogna escludere ogni ritorno, sotto qualsiasi forma, di classi e scuole speciali. Da anni il volontariato, soprattutto delle famiglie, ha aperto la strada alla società e alle istituzioni. Ha rotto il muro che le separava da una zona della vita, percorsa come altre, dal buio del dolore e dalla luce del risveglio. La federazione delle tre associazioni nazionali dell'autismo, che si chiama FANTASiA, ed altre associazioni che sono nate sul territorio, come AutAut di Reggio Emilia, chiedono strategie specifiche e metodologie avanzate di intervento, chiedono risorse adeguate, stabilità del personale della scuola. Ad esse oggi vanno date le risposte che da un Paese civile attendono: dunque, che l'Italia sia all'altezza almeno dei livelli della ricerca scientifica, dell'elaborazione culturale e pedagogica, dell'impegno sociale che tanti soggetti, singoli e associati, pubblici e privati, hanno raggiunto con le sole forze dell'umanità, della competenza, della passione civile. Che le istituzioni rispondano dunque con tempestività, con organicità, con forte solidarietà perché il Paese cresca in civiltà e l'Italia torni ad essere leader in Europa e nel mondo

Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, desidero consegnare il mio intervento, anche per la competenza degli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, che pure alcune note polemiche che non c'entravano molto con l'argomento. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno voluto sottoporre all'attenzione di questa Aula un problema così importante che si sta estendendo nell'arco degli anni spesso le nostre famiglie e i nostri bambini. Ringrazio il Governo per la sensibilità che dimostrerà nell'accogliere questa mozione.

Signor Presidente, onorevoli senatori, in merito alla mozione in esame, a cui si risponde per delega della Presidenza dei Consiglio dei ministri, prima di entrare nel vivo delle questioni poste al Governo, mi preme sottolineare che il tema oggetto della mozione è già all'attenzione del Ministero della salute e pertanto esprimo vivo apprezzamento per le finalità della mozione stessa e per gli argomenti sollevati. Prima di esprimere la posizione sugli impegni specifici sottoposti al Governo, ritengo necessario indicare i seguenti elementi valutativi. La natura e la complessità dei disturbi dello spettro autistico (DSA) impongono al Sistema sanitario nazionale, nelle sue articolazioni regionali che ne hanno specifica competenza organizzativa e gestionale, una serie di questioni in termini di riorganizzazione dei servizi per la messa in atto di protocolli adeguati ed aggiornati in termini di diagnosi precoce, di presa in carico del soggetto autistico attraverso un progetto riabilitativo multidisciplinare ed individualizzato, anche rispetto all'estrema variabilità soggettiva relativa ad ogni paziente. La continuità tra la diagnosi e l'impostazione di un adeguato progetto terapeutico integrato coinvolge inoltre la necessità assoluta di una serie di controlli periodici che verifichino gli effetti sul paziente con il pieno coinvolgimento della famiglia, della scuola o dei centri eventualmente frequentati al fine di monitorare costantemente lo stato di salute e di benessere generale della persona con autismo. Nonostante purtroppo una eziopatogenesi ancora incerta dei disturbi di tipo autistico, lo stato della ricerca a livello internazionale e dell'avanzamento delle conoscenze scientifiche sull'argomento sono all'attenzione di questo Ministero e devono vedere coinvolti anche gli assessorati regionali al fine di meglio organizzare la risposta territoriale, fondamentale per un corretto approccio alla patologia, anche in termini di assolvimento a quanto disposto in materia di livelli essenziali di assistenza e di una corretta gestione delle risorse umane, strutturali e finanziarie. In tal senso, ed in qualità di Sottosegretario per la salute con delega alla riabilitazione, mi preme sottolineare che, dopo adeguato percorso di confronto con le Regioni, le società scientifiche, i professionisti e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, il Ministero ha emanato le nuove linee guida sulla riabilitazione («Piano di indirizzo per la riabilitazione»), approvate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attraverso l'accordo del 10 febbraio 2011, che rappresentano una pietra miliare ed un punto di riferimento programmatico insostituibile al fine di determinare un corretto approccio, sia organizzativo che gestionale, per la definizione dell'offerta riabilitativa sul territorio nazionale. In questo senso, nella disamina del quadro attuale sono emerse numerose differenze territoriali rispetto ai migliori modelli e le migliori prassi attualmente acquisiti nei protocolli per un trattamento adeguato delle patologie e dei disturbi che necessitano di intervento riabilitativo. Sottolineo che la mia attenzione è puntata a quelle Regioni sottoposte a piani di rientro dal deficit affinché, nella loro necessaria attività di razionalizzazione, non determino ulteriori drammatici abbassamenti dell'offerta riabilitativa che, per una serie di svariati motivi, rappresenta oggi una emergenza della nostra epoca. Nel 2007, il Ministero della salute aveva avviato un Tavolo di lavoro sull'autismo, con l'obiettivo di stabilire un raccordo stabile tra Ministero, istituzioni coinvolte ed associazioni. Proprio a seguito delle raccomandazioni del Tavolo, e su sollecitazione delle società scientifiche di riferimento (Società italiana di neuropsichiatria infantile e Società italiana di psichiatria) e delle associazioni dei familiari, il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità hanno promosso una serie di attività di ricerca di base e clinica, quali la definizione di linee guida condivise e basate sull'evidenza per il trattamento delle sindromi autistiche, attualmente ancora in corso di stesura definitiva, che mi impegno a far approvare in tempi brevissimi; studi sulla componente genetica dei disturbi autistici e sulla valutazione del carico familiare; attività di ricerca di base in collaborazione con reti europee e con il *National Institute of Mental Health* statunitense, mirate soprattutto a comprendere il ruolo di potenziali geni coinvolti nelle sindromi autistiche in modelli sperimentali, al fine di individuare strumenti terapeutici innovativi. L'Istituto superiore di sanità ha avviato, in collaborazione con alcuni Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di neuropsichiatria infantile, una ricerca per l'individuazione di marcatori comportamentali e biologici del disturbo autistico già in fase neonatale, mediante strumenti di indagine non invasivi. Ricordo inoltre che, a cura dell'Istituto stesso, è attivo dal 25 maggio uno specifico sito *web* dedicato ai disturbi dello spettro autistico. Il sito tematico costituisce uno strumento a disposizione delle famiglie, degli operatori sanitari e degli educatori per ottenere informazioni aggiornate e controllate sulle evidenze scientifiche e cliniche e sulle ricerche attive in materia di autismo in Italia e nel resto del mondo. Il sito fornisce informazioni sulle linee guida nazionali e internazionali dedicate ai disturbi dello spettro autistico e contiene una sezione specifica, in continuo aggiornamento, rivolta principalmente alle famiglie, che possono accedere alle informazioni, suddivise per ciascuna Regione, riguardanti i centri e i servizi per la diagnosi e la presa in carico dei pazienti con autismo. Si condivide certamente l'importanza dell'istituzione di un Registro nazionale sui disturbi di tipo autistico al fine di consentire per questa specifica patologia la stima dell'incidenza e della prevalenza, nonché la valutazione dello stato e dell'organizzazione dei servizi per la diagnosi, la presa in carico sul territorio nazionale e del loro impatto. A tale proposito, si segnala che l'Istituto superiore di sanità ha presentato, congiuntamente con le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, nell'ambito del bando di ricerca finalizzata del Ministero della salute, un progetto sperimentale in tal senso tale da consentire l'avvio di un Registro pilota da estendere poi a tutte le Regioni. Inoltre, in merito alla promozione di forme di coordinamento e collaborazione tra le istituzioni interessate, al fine di sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale delle persone con autismo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha segnalato lo sviluppo di una serie di iniziative collegate alla realizzazione di attività a favore dell'autismo. Con la realizzazione del progetto nazionale "I Care" e con il progetto "Nuove tecnologie e disabilità" sono stati promossi e resi disponibili alle istituzioni scolastiche alcuni interventi innovativi per supportare i bambini con autismo. L'orientamento risiede nella visione unitaria di un quadro di integrazione scolastica dello studente disabile che comporta la valorizzazione delle potenzialità residue dell'alunno e del contesto sociale e culturale ai fini dell'inclusione della persona e della sua possibilità di un progetto di vita. Il MIUR, inoltre, nell'ottica della valorizzazione del territorio per il superamento delle disabilità, dal 2006 ha già istituito, con le azioni 4 e 5 del citato progetto, 98 centri territoriali di supporto dedicati all'uso ed alla promozione sul territorio per l'ampliamento delle potenzialità di apprendimento degli studenti mediante tecnologie educative per l'integrazione. Per quanto riguarda gli interventi rivolti ai familiari, dal punto di vista del sostegno, dell'informazione e della formazione, ne specifico la competenza strettamente regionale. Sottolineo altresì che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, per quanto di competenza, nel 2010 ha condotto un'indagine in collaborazione con le principali associazioni che seguono bambini ed adulti affetti da autismo al fine di comprenderne meglio il modello di lavoro, l'approccio terapeutico e il tipo di supporto fornito alle famiglie. Da ultimo, in merito agli impegni relativi all'implementazione di programmi di *screening* che favoriscano la diagnosi precoce attraverso il coinvolgimento dei pediatri di base e la promozione di processi di inclusione scolastica e sociale delle persone con autismo, anticipo che il Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha programmato due iniziative formative: un corso diretto ai pediatri di famiglia per informare sugli strumenti diagnostici e di *screening* precoce, al fine di favorirne la diffusione (previsto per novembre 2011), e un convegno indirizzato agli insegnanti, incentrato sugli interventi educativi e riabilitativi da applicarsi nel contesto scolastico con bambini con DSA. Alla luce delle valutazioni formulate, si esprime la posizione favorevole in ordine agli impegni contenuti nella mozione in esame si conferma l'impegno del Ministero della salute a sostenere le attività già avviate con il supporto dell'Istituto superiore di sanità e a promuovere ulteriori attività di ricerca di base, clinica ed epidemiologica, fondamentali per rispondere all'emergenza di salute rappresentata dai disturbi di tipo autistico.

testo scritto della mia dichiarazione di voto, vorrei sollecitare il Governo ad attuare le linee guida elaborate nel 2008 dal Tavolo nazionale di lavoro sull'autismo, istituito

Signor Presidente, abbiamo ascoltato l'intervento della Sottosegretaria, e capiamo che dobbiamo chiudere in fretta, però non mi pareva che questo fosse un argomento da liquidare così

offrire i servizi fondamentali a tutti i cittadini, in tutte le Regioni del Paese: soltanto così potremo continuare a parlare di Sistema sanitario nazionale.

che sta a cuore a noi della Lega Nord. In modo particolare, vogliamo far presente all'Assemblea e al sottosegretario onorevole Martini che ci si deve impegnare per fare in modo che agli studenti autistici venga garantita la continuità didattica dell'insegnante di sostegno, almeno per ogni ordine di scuola, e che l'insegnante di sostegno venga formato proprio per fare l'educatore di questi ragazzi particolari. Non ha senso aiutare un bambino autistico a trovare una via comunicativa con l'esterno per facilitargli la socializzazione e, nel contempo, cambiargli tutti gli anni l'insegnante di sostegno. So, per mia esperienza personale, che ci sono bambini autistici che non parlano e che comunicano solo attraverso il metodo della comunicazione facilitata: cambiare ogni anno l'insegnante di sostegno per questi bambini significa ricominciare ogni volta tutto daccapo proprio sul fronte della comunicazione, quello stesso fronte in cui si concentrano i disturbi dello spettro autistico. Voglio ringraziare la senatrice Biondelli e i colleghi senatori che hanno, attraverso questa mozione, messo in evidenza in maniera chiara, semplice ma importante le problematiche di questi ragazzi

tempestività dell'approvazione. Per questa ragione, la collega Biondelli ha giustamente deciso che rinunciassimo a lunghe dichiarazioni di voto. Tutto questo mi impedisce però di replicare, seppur brevemente, a qualche affermazione della collega Aderenti, della quale certamente rilevo la perfetta buona fede, con particolare riguardo alle questioni relative agli insegnanti di sostegno, al continuo cambio dei docenti e alla mancanza di una continuità didattica e formativa, che avrebbe costituito spunto del mio approfondimento che, come d'intesa, rassegno all'Aula per gli atti. Vorrei comunque esprimere un particolare apprezzamento per la collega Biondelli, alla cui sensibilità

ma un punto di partenza, anche per qualche questione che la Sottosegretario ha accennato, relativamente alla necessità che le Regioni omogeneizzino i propri interventi sui territori in maniera tale che non ci siano difformità da un territorio all'altro e da una Regione all'altra del nostro Paese. Non è un punto di arrivo, quello un punto di arrivo, quello di oggi, ma un punto di partenza, ed auspico, anzi, che questo ramo del Parlamento sappia far nascere un'iniziativa che sia più costante nel contatto con il mondo associativo del volontariato, con le famiglie che soffrono direttamente questo problema, con le attività dei formatori e con il Governo, in modo che si addivenga in tempi rapidi ad un più compiuto strumento legislativo, attingendo proprio all'esperienza di queste straordinarie realtà che operano sul territorio, spesso in ruolo di supplenza rispetto alle troppe latitanze delle istituzioni. Il voto del Gruppo del Partito Democratico sarà naturalmente favorevole.

vengono presentate mozioni, il Governo è d'accordo, si trova un consenso, ma poi alle mozioni non segue nulla. Siccome è un argomento delicato, di notevole importanza e l'intervento del Sottosegretario è stato illuminante rispetto alla questione,

Per essere persona di scuola, che ha vissuto per 35 anni, e forse anche di più, l'esperienza del contatto diretto con i portatori di handicap, in particolare per il mondo autistico, parliamo, e forse recepiamo, delle poesie ma non entriamo nel merito vero del problema. Le Regioni non sono in grado, a parte le linee guida, di affrontare il problema, soprattutto a livello di precauzione, che è quello che questa mozione vuole mettere in evidenza. La diagnosi precoce è una precauzione, che ritengo sia l'obbligo fondamentale per fare un'azione positiva nei confronti di questa realtà e di questo mondo. Signora Sottosegretario, la medicina scolastica non esiste.

indicazioni che siano cogenti per le Regioni e cogenti per le scuole, e di indicazioni che siano concertate a livello interministeriale, della sanità e dell'istruzione. Diversamente, infatti, non potremmo fare nient'altro che un discorso di assistenza del tutto generico, che non risolve il problema.

presentata da me e da molti altri colleghi del Partito Democratico in merito alla nota vicenda del batterio *killer* che ha contaminato determinate verdure, colpendo e provocando la morte di 17 sette cittadini europei. La rapida diffusione del batterio e le incertezze sulle modalità del contagio stanno allarmando i cittadini italiani, benché in Italia non siano stati registrati casi di contagio. Vorrei ricordare ai colleghi che in pochi giorni l'allarme sulla diffusione del contagio ha creato un danno economico al settore agricolo di circa 5 miliardi di euro, e sta mettendo in ginocchio tutto il settore orticolo. Per tali ragioni, chiediamo una immediata risposta in Aula dei Ministri in indirizzo per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per garantire la prevenzione del contagio dei cittadini italiani e quali misure siano state predisposte per far fronte all'emergenza legata alla diffusione del batterio in Italia.

perché ormai tutti gli allarmi alimentari in Italia sono la constatazione di fatto che la mancata attivazione dell'Agenzia fa fa dell'Italia l'anello debole della catena europea di controllo e prevenzione del rischio alimentare, con grave danno dei produttori agricoli e dei consumatori, che devono essere tutelati e tranquillizzati da eventuali rischi. *(Applausi

ai pochi colleghi ancora rimasti, che se esiste qualcuno che fa delle dichiarazioni di voto finale non leggendo un documento, quando interviene

nella qualità del dibattito), in questo modo si limita in maniera totale la possibilità, per il senatore che non legge, di poter sviluppare le proprie argomentazioni, perché non ha niente da considerare. Anche agli atti, pertanto, rimarrebbe un desiderio di possibilità. Non avendo noi un calendario particolarmente oberato di impegni, se non c'è neanche la disponibilità del Governo ad essere presente in questo breve dibattito, allora tanto vale rimandare, visto e considerato che si tratta di una discussione su mozioni e non su disegni di legge.